L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

di discussione del disegno di legge recante: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017";

il conto consuntivo del bilancio e il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, nonché i conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni statali dotate di autonomia. La proposta di bilancio a legislazione vigente per il 2018 assumerà, tra l'altro, come base di riferimento per la valutazione dei residui passivi, le risultanze definitive contenute nel rendiconto 2016, le quali sono altresì evidenziate nel disegno di legge di assestamento per il 2017, che verrà poi illustrato, ai fini della determinazione degli eventuali adeguamenti delle autorizzazioni di pagamento. È allegato al disegno di legge il rendiconto economico, che espone le risultanze economiche per ciascun Ministero e i prospetti di riconciliazione con le risultanze del rendiconto finanziario. Inoltre, è allegata l'illustrazione delle risultanze delle spese relative ai programmi aventi natura o contenuti ambientali, allo scopo di evidenziare le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente. Grazie alle innovazioni apportate alla legge di contabilità con l'aggiunta dell'articolo 47-*bis* da parte del decreto legislativo n. 93 del 2016, al presente rendiconto sono allegate anche indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla Tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Con riferimento ai risultati della gestione di competenza, nell'insieme, si registra un miglioramento dei saldi sia rispetto alle previsioni definitive, come risultanti dalla legge di assestamento 2016, sia rispetto ai risultati conseguiti nell'esercizio 2015. In particolare, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2016 presenta un valore negativo pari a 11,1 miliardi di euro, con un miglioramento di ben 30,4 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2015, che si era, invece, assestato a un valore negativo di 41,5 miliardi. Rispetto alle previsioni definitive, tale saldo è risultato migliore di 27,8 miliardi, 27,8 miliardi, posto che era previsto attestarsi, nel 2016, a un valore negativo di 38,9 miliardi di euro. Oggettivamente c'è stato un miglioramento non indifferente. L'avanzo primario

Il saldo delle operazioni correnti (risparmio pubblico) nel 2016 è risultato pari a 27,8 milioni di euro. Si evidenzia un miglioramento di 36,9 milioni rispetto al 2015,

Il ricorso al mercato (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si è, infine, attestato nel 2016 ad un valore pari a meno 207,1 miliardi di euro. Anche tale saldo è in miglioramento rispetto al 2015, attestandosi a un valore più basso di circa 50 miliardi. L'entità complessiva degli accertamenti di entrata, comprensivi delle entrate per accensione di prestiti, pari a 845,9 miliardi 845,9 miliardi di euro, evidenzia un andamento positivo rispetto all'anno precedente (16,8 miliardi euro, che rappresenta circa il 2 per cento). Tale aumento è il frutto dell'incremento delle entrate correnti, pari a 16,7 miliardi, mentre la diminuzione delle entrate di alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti,

ammontano a 788,4 miliardi e presentano, rispetto ai risultati dell'anno precedente, una riduzione complessiva degli impegni di spesa di 38,2 miliardi di euro. C'è, quindi, un calo del 4,6 Per ciò che attiene alla spesa corrente, gli impegni sono stati pari a 549,6 miliardi di euro, con una diminuzione rispetto all'anno precedente di 20,1 miliardi, pari al 3,5 Per le spese in conto capitale, con impegni pari a 42,8 miliardi, il rendiconto 2016 segnala un lieve aumento rispetto all'anno precedente 1,5 miliardi (3,6 per cento). Tuttavia, si tratta di un ammontare ben lontano da quello raggiunto in altri esercizi, come ad esempio nel 2014, anno in cui le spese in conto capitale avevano raggiunto i 76,8 miliardi. Guardando la serie storica dal 2008, l'anno in esame è stato infatti quello con la spesa in conto capitale più bassa dopo il 2015. E questo è un elemento su cui il Governo deve

Il peso della spesa complessiva, in rapporto al PIL, è diminuito dal 50,24 per cento del PIL nel 2015 al 47,14 per cento Passando poi alla gestione dei residui, l'entità degli stessi nell'esercizio 2016 è rimasta su livelli considerevoli, anche per effetto delle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. che hanno previsto l'aumento del termine di conservazione dei residui di spese in conto capitale e dei trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, portandoli da due a tre anni. Inoltre, si prevede non più l'automatica perenzione dei residui passivi di parte corrente dopo due anni, ma un'attività di riaccertamento da parte delle amministrazioni. In sintesi, il conto dei residui al 31 dicembre 2016 espone residui attivi per 212,2 miliardi di euro e residui passivi per 134,4 miliardi di euro, con un'eccedenza attiva di 77,8 miliardi di euro. I residui attivi sono aumentati di circa 4 miliardi (quasi il 2 per cento in più) rispetto al 2015, mentre l'incremento dei residui passivi è stato di circa 21,4 miliardi (pari al 18,9 In particolare, l'incremento dei residui attivi complessivi è legato non a quelli di nuova formazione, che si sono ridotti di 4,7 miliardi, ma a quelli provenienti da esercizi precedenti, aumentati di 8,7 miliardi. Anche l'incremento dei residui passivi è ascrivibile non a quelli di nuova formazione, che rimangono stabili a circa 66 miliardi, ma alla notevole diminuzione delle perenzioni che, per effetto delle modifiche normative citate, sono diminuite dell'86 Sono stati infatti circa 16,4 miliardi i residui passivi mantenuti, che sarebbero andati in perenzione se non vi fosse stato l'allungamento di un anno del periodo di conservazione in bilancio. Nel rendiconto sono poi esposte e illustrate le risultanze della gestione di cassa: va ricordato in proposito che la gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. La gestione di cassa presenta, sotto un profilo generale, un andamento analogo a quella di competenza, con un miglioramento sia rispetto alle previsioni definitive sia rispetto ai risultati conseguiti nel 2015. Il conto generale del patrimonio evidenzia una eccedenza passiva di 1.798 miliardi, con un peggioramento di circa 39,6 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2015, dovuto a un aumento delle passività (circa 63,9 miliardi) solo in parte compensato dall'incremento delle attività (aumentate di 24,4 miliardi). In particolare, il totale delle attività ammonta a 987 miliardi di euro, di cui 675,9 miliardi di attività finanziarie (in aumento di 18,8 miliardi rispetto al 2015); 306,8 miliardi di attività non finanziarie prodotte, che comprendono beni materiali e immateriali prodotti, materie prime e prodotti intermedi, prodotti finiti, oggetti di valore e d'arte (beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi), in aumento di 5,5 miliardi rispetto al 2015; 4,2 miliardi di attività non finanziarie non prodotte, che comprendono i beni materiali non prodotti, ossia terreni, giacimenti e risorse biologiche non coltivate Il totale delle passività ammonta a 2.785 miliardi circa e si riferisce interamente a passività di natura finanziaria. Questo è il peso che ha, Il giudizio di parificazione da parte della Corte dei conti ha rilevato alcune irregolarità elencate nell'apposito referto trasmesso al Parlamento. In particolare, la Corte dei conti ha rilevato, nella decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle entrate, entrate, dei capitoli e articoli per i quali sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel rendiconto e quelli dei conti periodici delle amministrazioni; dei capitoli e articoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto in rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo. Per superare tali discordanze, il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha avviato diverse attività anche con gli uffici territoriali che seguono la gestione di diverse entrate erariali, volte a migliorare la rappresentazione delle risultanze gestionali e, conseguentemente, a limitare gli interventi di rettifica operati in sede di predisposizione del rendiconto (come, ad esempio, la procedura di compensazione per l'eliminazione dei residui attivi che presentano segni negativi). Segnalo, altresì, che c'è un continuo confronto sul piano tecnico tra la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti volto ad approfondire gradatamente le specifiche problematiche più volte segnalate dalla Corte stessa. Per quanta riguarda i resti da versare in conto residui, la Corte rileva l'aumento registrato nel 2016 rispetto al 2015. A questo proposito, si fa presente che gli aumenti sono in via di riassorbimento e saranno oggetto di regolazione contabile nell'esercizio in corso. Sul versante della spesa, invece, la Corte ha rilevato le irregolarità dei capitoli che presentano eccedenze nei conti della competenza, dei residui e della cassa, concernenti tutte le amministrazioni dello Stato, ad eccezione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La nota del dipartimento precisa che le eccedenze che si generano a livello di capitolo di spesa trovano compensazione con le economie registrate all'interno dell'unità di voto di appartenenza. Si fa presente che un articolo specifico del disegno di legge di approvazione del rendiconto è dedicato a proporre una sanatoria legislativa per gli eccessi di spesa (le eccedenze, appunto) rispetto agli stanziamenti definitivi eventualmente verificatisi in ciascuna unità di voto, qualora non siano compensate dalle economie realizzate all'interno dell'unità di voto stessa. Le eccedenze registrate riguardano essenzialmente spese fisse (stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi del personale, compresi oneri sociali e IRAP), i cui pagamenti vengono eseguiti con modalità del tutto particolari previste dalla legge di contabilità (nella quasi totalità dei casi mediante l'esecuzione di ruoli di spesa fissa). Hanno una articolazione temporanea rigida, per cui la contabilizzazione avviene solo dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, generando un esubero di impegno/pagamento rispetto alle previsioni, con il conseguente formarsi delle eccedenze. L'inderogabilità e l'indifferibilità delle spese stesse comportano, del resto, la imprescindibilità della loro erogazione e, quindi, il verificarsi dell'eccedenza. In merito all'andamento dei residui passivi per il 2016, si fa presente che le novità introdotte dal decreto legislativo n. 83 del 2016 (cioè la riforma del bilancio) hanno influenzato tale andamento. L'articolo 6 del citato decreto ha modificato la normativa relativa al regime contabile dei residui passivi, con particolare riferimento alla disciplina della conservazione dei residui di bilancio, nonché alle attività di accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi di bilancio e dei residui passivi perenti; per cui si giustifica l'andamento del 2016 non in linea con quello del 2015. Sul piano del patrimonio, l'organo di controllo ha rilevato discordanze e omissioni sui beni immobili dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti; i beni mobili di otto Ministeri; i residui attivi e passivi delle poste del Ministero dell'economia; il fondo scorta del Ministero della difesa; i crediti concessi ad enti pubblici e ad istituti di credito del Ministero dell'economia. Le discordanze e omissioni rilevate dalla Corte dei conti derivano dalle difficoltà riscontrate nell'integrazione dei sistemi informatici. Le istituzioni interessate stanno lavorando per risolverle, visti i rilievi. Infine, in merito alle osservazioni della Corte in materia di conto del patrimonio, la nota della Ragioneria rileva che non è stata ancora adottata la classificazione Sec 2010. L'applicazione è stata rinviata nel tempo per motivi di economicità ed efficienza. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti

atto del fatto che sicuramente molte politiche da noi approvate e proposte dal Governo incominciano a dare i loro frutti e penso sia opportuno sottolinearlo.

2875*. Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghe e colleghi, il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 consta di tre articoli ed è corredato di tabelle con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, suddivisi per Dicasteri e amministrazioni autonome. Il disegno di legge in esame è il primo a essere predisposto conformemente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 90 del 2016

Con le modifiche qui ricordate, sono stati messi a regime i margini di flessibilità concessi alle amministrazioni ed è stato previsto il rispetto di un vincolo sul saldo del bilancio di cassa programmatico, che si aggiunge a quello di competenza. Il testo è stato corredato di una relazione tecnica che illustra la coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. È stato inoltre previsto che la relazione tecnica analizzi gli effetti delle principali variazioni proposte al bilancio dello Stato e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Resta immutata la natura di legge formale dell'assestamento, in quanto le previsioni di bilancio in essa contenute devono essere formulate a legislazione vigente. Per quanto riguarda il complesso delle variazioni derivanti da atti amministrativi e proposte nel disegno di legge in esame, si determina un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari a circa 56 miliardi di euro,

Con riferimento invece al bilancio di cassa, il peggioramento del saldo ammonta a circa 20 miliardi di euro, con un saldo netto da finanziare che passa da 102,6 miliardi a 122,6 miliardi. ciò è imputabile a variazioni per atti amministrativi pari a meno 21,9 miliardi per quanto riguarda la competenza e a meno 21,8 miliardi per la cassa, che sono solo parzialmente compensate nelle proposte di assestamento con effetti migliorativi pari rispettivamente a circa 4,5 e 1,8 miliardi di euro. Per completezza d'informazione va segnalato che, dal lato delle entrate, le proposte di variazioni comportano un miglioramento dell'indebitamento netto pari a circa un miliardo di euro, però vengono compensate dal lato delle spese da un peggioramento di pari ammontare, così da determinare un effetto complessivo nullo. Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2017, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2017 - espressi in termini di competenza e considerati al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA - evidenziano un miglioramento del solo risparmio pubblico e un peggioramento del saldo netto da finanziare, del ricorso al mercato e dell'avanzo primario. Il saldo netto da finanziare (corrisponde alla differenza tra entrate finali e spese finali) presenta una variazione di segno negativo pari nel complesso a 17,4 miliardi, un valore comunque coerente con il limite massimo stabilito dall'allegato 1 della legge di bilancio per il 2017, come successivamente modificato. La previsione assestata del saldo è determinata dal peggioramento per 21,9 miliardi per atti amministrativi e dal miglioramento per 4,5 miliardi per le proposte formulate dal disegno di legge in esame. Quest'ultima categoria è il risultato dell'aumento delle entrate per 2,8 miliardi e della riduzione della spesa per interessi per 1,9 miliardi, in parte compensate dall'aumento delle spese correnti e in conto capitale per circa 300 milioni di euro. Con riferimento al risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi), le previsioni assestate migliorano, rispetto a quelle iniziali, per un valore di 2,9 miliardi. I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti)

Un dato da sottolineare è il sensibile peggioramento dell'avanzo primario che, nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle assestate, subisce un dimezzamento, portandosi a poco più di 19,3 miliardi di euro. Per quanto riguarda le entrate finali, le previsioni assestate aumentano di 5,3 miliardi rispetto a quelle iniziali, come risultato di un incremento delle entrate tributarie per 1,8 miliardi e di quelle extratributarie per 3,5 miliardi. Le previsioni assestate delle spese finali fanno registrare un incremento di 22,7 miliardi. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, dal lato delle entrate tributarie si registrano variazioni in aumento per circa 370 milioni di euro. Sul fronte delle entrate extratributarie si registrano variazioni in aumento per poco più di 2,1 miliardi, che sono quasi esclusivamente riferibili all'applicazione di provvedimenti successivi alla legge di bilancio, di cui 2 miliardi imputabili all'attuazione dell'articolo 1, comma 433, della medesima legge di bilancio, che ha previsto il versamento all'entrata - per alimentare il Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali - dei residui relativi alle anticipazioni alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e delle somme disponibili sulla contabilità speciale istituita per la ristrutturazione del debito regionale. Le variazioni per atto amministrativo hanno incrementato la spesa di 24,4 miliardi quale somma di 4,1 miliardi di maggiori spese correnti e 20,3 miliardi di spese in conto capitale. L'incremento delle spese correnti è imputabile alle variazioni relative ai redditi da lavoro dipendente (1,8 miliardi) per riassegnazioni delle somme relative delle competenze accessorie del personale che erano state versate a fine 2016 e ai trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche per l'attribuzione di circa 900 milioni di euro al Fondo per la reiscrizione dei residui di parte corrente e di circa 100 milioni per trasferimenti ai Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale. L'aumento della spesa in conto capitale (pari a 20,3 miliardi) è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 237 del 2016 (il cosiddetto decreto salva-risparmio), che ha comportato un incremento delle acquisizioni di attività finanziarie per 20 miliardi, un incremento dei contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche per 215 milioni e degli investimenti fissi lordi per 146 milioni, oltre che minori trasferimenti in conto capitale per circa 190 milioni. Le proposte di assestamento formulate con il disegno di legge in esame migliorano i saldi di finanza pubblica sia aumentando le entrate (più 2,8 miliardi), sia riducendo le spese finali (meno 1,6 miliardi) e il rimborso delle passività finanziarie (meno 5 miliardi). Con riferimento alle spese finali la riduzione di 1,65 miliardi è imputabile alla consistente riduzione della spesa per interessi pari a 1,95 miliardi di euro (somma di 1,15 miliardi per la dinamica dei tassi di interesse e di 0,8 miliardi per minori interessi sui conti correnti di tesoreria), che quindi attenua l'aumento di 253 milioni della spesa corrente al netto degli interessi e di 45 milioni della spesa in conto capitale; all'interno di queste ultime voci si segnalano le seguenti variazioni. In primo luogo, le variazioni delle autorizzazioni di cassa comportano, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento di tutti i saldi ad eccezione del risparmio pubblico. L'entità del peggioramento del saldo netto da finanziare è di circa 20 miliardi, mentre la necessità di ricorrere al mercato registra un incremento di 15,2 miliardi, raggiungendo l'importo di quasi 372 372 miliardi; l'avanzo primario, partendo dal valore negativo di quasi 23,4 miliardi, giunge a un importo ugualmente negativo di poco meno di 45,7 miliardi, con un peggioramento percentuale di poco inferiore al 96 per cento. Il solo risparmio pubblico migliora di 3,3 miliardi passando da circa 61,2 miliardi a 57,9 miliardi. Degna di nota è invece la differenza di quasi 2,7 miliardi di euro tra la consistenza delle spese finali in termini di competenza e di quelle in termini di cassa, spiegata dallo smaltimento dei residui passivi. In particolare, con riferimento alle spese in conto capitale, queste registrano un incremento solo di 45 milioni con riferimento agli stanziamenti di competenza e di quasi 2,5 miliardi in termini di cassa, a causa delle variazioni proposte in relazione alla effettiva consistenza dei residui passivi di conto capitale, che pesano sulla voce in termini di cassa, e il cui pagamento è già considerato nelle stime tendenziali di finanza pubblica. Per quanto riguarda invece le spese di parte corrente, al fine di smaltire i residui di parte corrente, vengono avanzate proposte di integrazione delle dotazioni di cassa che spiegano la differenza tra queste ultime e le corrispondenti proposte di assestamento in termini di competenza. Vi sono poi una serie di proposte di assestamento che riguardano le missioni. La composizione delle variazioni formulate dall'assestamento, appunto articolate per missioni, mette in evidenza una serie di elementi, tra cui cito le variazioni più significative, innanzitutto, la minore necessità di rimborso di prestiti internazionali, con una riduzione della missione «Debito pubblico» pari a 6,15 miliardi in termini di competenza e 6,4 miliardi in termini di cassa. inoltre minori spese della missione «Politiche previdenziali» per 1,2 miliardi di euro (competenza e cassa), imputabili all'adeguamento dell'effettivo fabbisogno dell'INPS. La riduzione di spesa delle «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» pari a circa un miliardo in termini di competenza (841 milioni in termini di cassa), è dovuta principalmente alle minori regolazioni contabili delle entrate erariali riscosse dalle Regioni a Statuto speciale, con riferimento anche ad anni precedenti. Vi è poi l'aumento delle spese della missione «Politiche per il lavoro» per 1,4 miliardi in termini di competenza e 1,3 miliardi in termini di cassa, a causa dei maggiori oneri relativi ai trattamenti di CIG straordinaria e ai connessi trattamenti di fine rapporto. Cito poi l'incremento di 990 milioni (solo in termini di cassa) della missione «Soccorso civile» in seguito alle assegnazioni in favore degli uffici speciali all'Aquila e ai Comuni del cratere per la ricostruzione.

dei quali 66,1 miliardi di nuova formazione, cioè derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2016, mentre 67,9 miliardi provengono dagli esercizi precedenti. L'incremento di 24,4 miliardi dei residui passivi finali è imputabile all'aumento di quelli di parte corrente per 18,6 miliardi e di quelli di conto capitale per 5,8 miliardi. punto importante è la coerenza tra i saldi programmatici del bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico. La relazione tecnica fornisce a tal riguardo elementi circa la coerenza tra i saldi programmatici del bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nel Documento di economica e finanza (deliberato dal Consiglio dei ministri l'11 aprile 2017 e modificato dal provvedimento di assestamento del bilancio dello Stato) attraverso un prospetto di raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato-previsioni assestate e il conto della pubblica amministrazione programmatico assestato per il 2017. L'indebitamento netto del bilancio assestato riclassificato è pari a 34,8 miliardi di euro, quello associato al conto economico della pubblica amministrazione, comprensivo di previsioni assestate, è pari a 39,6 miliardi di euro e infine quello relativo al conto economico programmatico sempre della pubblica amministrazione, comprensivo di previsioni assestate e integrato

In particolare si segnala l'articolo 2 comma 1 che, modificando il comma 2 dell'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, aumenta a 79,5 miliardi di euro l'importo massimo di emissione di titoli pubblici in Italia e all'estero per l'anno 2017, al netto di quelli da rimborsare e per regolazioni debitorie, rispetto ai 59,5 miliardi previsti dalla legge di bilancio. Il comma 2, che modifica il comma 3 dell'articolo 3 della legge di bilancio per il 2017, in materia di quantificazione dell'importo massimo degli impegni assumibili dalla SACE dalla SACE SpA per l'anno finanziario 2017, opera un trasferimento di risorse dalle garanzie a breve durata a quelle a media e lunga durata. In particolare, vengono ridotte da 5 a 2 miliardi di euro le garanzie di durata fino a due anni e aumentate da 14 a 17 miliardi di euro le garanzie di durata superiori ai due anni. Infine, va menzionato l'articolo 3 del provvedimento, che corregge la denominazione del fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso incluso nello stato di previsione per l'anno finanziario 2017, finanziario 2017, trasformandola in fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso. Si prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, oltre a ripartire le risorse del fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, possa anche assegnare direttamente le medesime risorse all'istituto gestore della Tesoreria dello Stato anche in conto residui. Quest'ultimo, ai sensi della misura in oggetto e secondo lo schema trasmesso

perché credo sia importante inserire i dati di assestamento del bilancio di esercizio 2017 all'interno di un contesto che riguarda naturalmente il dato economico più rilevante di quest'anno, ovvero la conferma che la nostra economia è in crescita e che questa crescita si sta consolidando ed è in via di sensibile accelerazione.

si registra un miglioramento rispetto all'anno precedente, dovuto agli effetti della crescita economica, ma anche alle misure di consolidamento dei conti pubblici, tra cui la manovra correttiva definita prima dell'estate. Come più volte sottolineato, per la politica economica del nostro Paese è fondamentale riuscire a coniugare la più generale strategia di sostegno e rilancio della crescita con una riduzione del disavanzo pubblico e del rapporto tra debito e PIL,

il Ministro dell'economia e delle finanze e, in generale, il nostro Governo. Va detto che questa strategia del sentiero ha cominciato a dare i primi frutti positivi in particolare quest'anno. di risultati importanti che vanno sottolineati, anche se va aggiunto che la strada da percorrere per la politica economica del nostro Paese resta in qualche modo lunga e difficile, perché vogliamo che lo *stock* del debito pubblico non solo sia in diminuzione in rapporto al PIL, ma anche che venga riportato a dimensioni più che sostenibili, mantenendo allo stesso tempo una politica di sostegno alla ripresa.

un sentiero di crescita sostenuta, che segnala un aumento della dinamica di espansione rispetto all'anno precedente. Questa tendenza al miglioramento della congiuntura appare condivisa dalla maggior parte delle aree dell'economia mondiale ed è la prima volta da circa dieci anni. È evidente che il nostro Paese ha l'opportunità di proseguire e consolidare il proprio percorso di crescita ad un ritmo altrettanto sostenuto ed ancor più sostenuto di quello in corso. Questo naturalmente ci consentirà, altresì, di porre il rapporto tra debito e PIL su un sentiero significativamente discendente. quindi molto importanti le nostre scelte come Paese e nulla potremo ottenere se non manterremo una stabilità politica e se non continueremo a sviluppare e ad accelerare il processo di riforme interne. Concludo, quindi, dicendo che serve sostenere la ripresa economica, continuando a garantire il risanamento dei nostri conti pubblici, come abbiamo fatto in questi in questi anni e soprattutto nel periodo più recente, perché riteniamo che questa sia la sola strada che potrà aiutare il nostro Paese a cogliere questa opportunità di espansione per molti versi unica che si sta profilando a livello internazionale ed europeo.

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, l'assestamento 2017 e il rendiconto 2016 sono gli ultimi documenti che fotografano complessivamente, a consuntivo, la politica economica del centrosinistra in questi quattro anni. La maggioranza è la stessa e la compagine di Governo sostanzialmente la medesima, con lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze che ha determinato l'andamento dei conti pubblici, sia con il Governo Renzi che con quello Gentiloni. Ovviamente l'ex *premier* Renzi sta rivendicando in questi giorni i successi sulla base delle proiezioni del PIL, visto in crescita tendenziale all'1,5 per cento e sulla base dei dati ISTAT entrambi i dati sono poco lusinghieri se raffrontati con quelli degli altri Paesi europei, che hanno agganciato la ripresa internazionale con percentuali sulla crescita e sugli occupati di gran lunga superiori alle nostre e soprattutto se confrontati con i livelli pre-crisi. Ed ancora ci si sta chiedendo se questa debole ripresa sia ciclica o strutturale, quando in realtà è legata soprattutto a fattori esogeni. Il dato sul debito pubblico, ovviamente, non viene mai citato, ma è quello che avrà le maggiori ripercussioni sui conti pubblici, posto che ormai si è portato a ridosso dei 2.300 miliardi, dopo quattro anni di conti pubblici in *deficit*: 233 miliardi di debito in più di quando è cominciata l'avventura di questo Governo di centrosinistra, quasi 390 miliardi in più rispetto all'ultimo Governo di Silvio Berlusconi. Risultato: il milione di posti di lavoro reclamato da Renzi è largamente a tempo determinato, mentre sugli italiani, purtroppo, conteremo 2.300 miliardi di debito che sono a tempo indeterminato. I numeri che si porta dietro l'assestamento si ripercuoteranno sia sulla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza che sulla legge di bilancio per il 2018. I principali saldi di bilancio hanno valori negativi. Sale il saldo netto da finanziare di 17 miliardi. Scende l'avanzo primario di oltre 19 miliardi, fotografando la differenza tra entrate e spese finali, al netto degli interessi. Da rilevare che salgono sia le spese finali (quasi 23 miliardi) che le entrate finali per effetto di un aumento delle imposte e tasse per oltre cinque miliardi e questo non ci fa sicuramente piacere. Quest'ultima è una cifra che non può essere solo la risultante del debole incremento del PIL del 2017, né il risultato del contrasto all'evasione, ma segnala un vero e proprio aumento del prelievo fiscale. Le spese finali scendono grazie alla riduzione della spesa per interessi dovuta alle politiche monetarie della Banca centrale europea. Il fenomeno migratorio si mangia un altro mezzo miliardo, ulteriore rispetto alle previsioni iniziali di bilancio. Abbiamo provato a emendare le ricche poste riservate ai migranti, girandole a favore delle famiglie italiane, sempre più in difficoltà, considerato, oltretutto, che gran parte di questi soldi oltre ad alimentare un flusso per ora ridotto, ma non fermato, verso l'Italia, nutrono molte clientele e molto malaffare. Abbiamo, appunto, provato a spostare qualche soldo a favore delle famiglie e degli anziani, ma eravamo di fronte a un testo inemendabile. Inoltre, la spesa corrente sale ancora e questo è un indicatore assolutamente negativo, perché rimane anch'esso come lascito all'Esecutivo che verrà. Questo dato indica, inoltre, che poco si è fatto sul lato della *spending review* ed infatti cresce la spesa legata alle variazioni dei redditi da lavoro dipendente. Manca ancora, nonostante noi l'avessimo chiesta più volte, quella revisione delle piante organiche della pubblica amministrazione,

costretti a diminuire i servizi e gli investimenti sui territori di competenza, oltre che sugli enti di area vasta come le provincie, menomate ma mai abolite, che ritorneremo a finanziare poco nel 2018 e un po' di più nel 2019. Sostanzialmente ci

anche a livello centrale e delle società partecipate. Tra l'altro, sale la spesa per consumi intermedi, ma soltanto una cifra inferiore al mezzo miliardo è stata utilizzata per pagare i debiti pregressi maturati nei confronti delle imprese. Il prossimo Governo erediterà almeno (e dico almeno) 10 miliardi da saldare alle nostre aziende e su questo bisognerà arrivare a una soluzione per smaltire definitivamente l'arretrato certificato, avviandosi ad introdurre tempi europei per saldare chi fornisce beni e servizi al settore pubblico. Nell'economia reale bisogna continuare a fare investire i risparmiatori, considerato che le misure adottate funzionano (penso ad esempio ai PIR), agevolando ulteriormente ogni forma di investimento duratura. Questo è l'unico antidoto alle speculazioni finanziarie mordi e fuggi. Siamo assolutamente convinti che le agevolazioni al risparmio e agli investimenti possano determinare sulla crescita economica un effetto certamente superiore a quello che ha avuto la misura degli 80 euro. Ovviamente, la considerazione più importante è relativa al fatto che buona parte della ripresa è dovuta alla politica monetaria della BCE, così come il piano di acquisto di titoli di Stato ha regalato minori oneri sul debito pubblico e questo sicuramente fa bene ai conti dello Stato. Anche l'acquisto di *corporate bond* ha segnato un passo diretto della Banca centrale a supporto dell'economia reale. Quindi, siamo consapevoli che dopo le elezioni politiche, dovremo preoccuparci non tanto di chi sarà il nuovo Ministro dell'economia, ma di chi sarà il nuovo Governatore della Banca centrale europea perché possa proseguire quelle politiche che tanto ci hanno fatto bene in questi anni. Per concludere, tirate le somme dei numeri di questo rendiconto per il 2016 e di questo assestamento per il 2017, i documenti in esame segnalano soprattutto le politiche economiche "del rinvio" adottate in questi anni

L'annunciata manovra di 25 miliardi sembra essere inserita nello stesso solco di quelle che l'hanno preceduta, quindi non ci aspettiamo alcuna inversione di rotta che possa dare una mano al Paese. Il voto contrario dei senatori del Gruppo Forza Italia su questi conti pubblici è quindi serio, ponderato e convinto ma anche molto preoccupato.

abbiamo oggi al nostro esame il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato per il 2016 e il disegno di legge relativo alle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno 2017.

La legge stabilisce che tale documento dovrebbe essere presentato in Parlamento nel mese di giugno però è bene che l'Assemblea non venga a conoscenza di queste cose o ne venga a conoscenza solo relativamente perché i risultati sono talmente disastrosi che è meglio non renderli noti. Dunque se ne discute alla ripresa dei lavori, confidando nel fatto che nessuno abbia esaminato i documenti due documenti che fotografano le conseguenze dirette delle scelte economiche generali effettuate dal Governo negli anni precedenti. Non entrerò nel dettaglio della serie di rilievi critici sui due provvedimenti che sono stati sollevati dalla Corte dei conti, che nella relazione sul rendiconto 2016 ha riscontrato anomalie e incongruenze nella contabilità delle amministrazioni, costituite essenzialmente dalla rilevazione di capitoli nel "da riscuotere" e nel "da versare", sia nel conto di competenza che nel conto residui. Sono state poi riscontrate varie varie anomalie in tutta la contabilità. Tutto questo basterebbe per rimandare indietro il rendiconto generale e ricominciare da capo. Mi preme invece sottolineare quanto è successo in questo anno: il debito pubblico è aumentato di un'altra cinquantina di miliardi, 48 miliardi per la precisione. Rilevo come nel 2015 il debito pubblico era aumentato di 33,8 miliardi. Abbiamo avuto un incremento notevole del debito pubblico rispetto all'anno precedente. Sarà una congiuntura o sarà la situazione del momento, ma se andiamo a guardare uno spazio temporale di febbraio del 2012 e lo scorso mese di giugno, che è l'ultimo dato reso noto dalla Banca d'Italia, il debito pubblico è cresciuto di 353 miliardi. Negli ultimi cinque anni il debito pubblico ha avuto un incremento del 15 per cento. Se andiamo ancora più indietro e vediamo che cosa è successo dal Governo Monti in poi (governi appoggiati dal Partito Democratico), il risultato è ancora più clamoroso: 375 miliardi di incremento di debito pubblico. Governi nati per risanare il debito pubblico hanno condotto il Paese sull'orlo del baratro.

la Germania ha speso appena il 20,7 per cento, la Francia il 21,9 e il Regno Unito il 23,2.

Questo pone una serie di problemi, perché nei prossimi cinque anni, cioè nella prossima legislatura, il debito pubblico italiano da piazzare sarà di oltre mille miliardi, perché sono a scadenza titoli di Stato che in cinque anni equivalgono Il problema che si pone però è come questo maggiore debito pubblico viene utilizzato: se il debito pubblico è utilizzato per far crescere l'economia, migliora il rapporto debito-PIL e quindi può anche essere giustificato. Purtroppo in Italia questo aumento del debito pubblico non ha portato miglioramenti all'economia del Paese. Il PIL non cresce. Mentre gli altri Paesi europei hanno superato il livello di PIL che avevano nel 2008, prima della crisi, in Italia siamo a 6,5 punti percentuali rispetto al 2008. Ciò deriva dal fatto che ormai chiudono ogni anno centinaia di imprese. Negli ultimi otto anni si sono perse 158.000 imprese tra artigianato e commercio al dettaglio.

non possiamo dimenticare che da quell'anno a oggi la popolazione è aumentata di circa 900.000 unità. Dobbiamo allora guardare a un altro parametro: le unità di lavoro, l'indicatore della quantità di lavoro complessiva che ci dà un dato più realistico. nove anni fa abbiamo perso un milione di unità lavoro. È vero che il numero di occupati è tornato ai livelli del 2008, ma se uno lavora una settimana, uno o due mesi o un anno, non è un lavoro vero ed effettivo. Voi truccate le cifre da questo punto di vista e illudete gli italiani che sono aumentati i posti di lavoro. In realtà, abbiamo perso 350.000 posti di lavoro. Questo è il risultato delle vostre politiche

Invece, queste cose le chiudiamo in tre ore il giorno dopo la ripresa dei lavori; archiviamo il consuntivo; l'importante è che non se ne parli, perché i risultati sono davvero disastrosi.

Presidente, intervengo molto rapidamente perché la discussione ha sollevato pochi elementi problematici rispetto alle Mi pare sia utile semplicemente sottolineare un elemento: i dati del rendiconto e, in una certa misura, anche quelli dell'assestamento testimoniano la fecondità dell'approccio alle scelte fondamentali di politica fiscale messo in atto nel corso di questi anni. La metafora, cui anche io faccio ricorso, è quella spesso usata dal Ministro dell'economia del nostro Paese relativa al cosiddetto sentiero stretto che il nostro Paese deve essere in grado, con la sua politica economica e fiscale, di percorrere tra due esigenze entrambe assolutamente rilevanti. rispetto ad altri Paesi europei, più forti esigenze di consolidamento fiscale, anche quando, come sta accadendo, gli orientamenti di politica economica e fiscale in sede comunitaria tendono a diventare più favorevoli rispetto al perseguimento di obiettivi di crescita e a discostarsi dalla univocità del riferimento alle esigenze di consolidamento, che ha caratterizzato la fase precedente degli orientamenti di politica fiscale dell'Unione europea. Quindi, anche quando questo mutamento avviene, nel caso italiano, l'esigenza di consolidamento, sotto il profilo fiscale, è assolutamente ancora forte. Ciò perché il volume globale del debito pubblico che abbiamo accumulato è decisamente più grande rispetto a quello degli altri grandi *partner* dell'Unione monetaria. Questo elemento elemento ci spinge a mantenere avanzi primari relativamente grandi a paragone di quelli di altri Paesi e ci spinge ad orientarci nel sostegno alla crescita e nell'affrontare i problemi dell'eccesso di disuguaglianza, che caratterizzano il nostro Paese, in una chiave nella quale dobbiamo sempre tenere in conto l'esigenza di non travolgere i risultati che abbiamo ottenuto sul versante della stabilità finanziaria. che nel corso di questi anni si è dimostrato che il Governo ha saputo tenere conto - questo dicono i numeri ad oggi - anche dell'esigenza di abbinare alle scelte orientate all'obiettivo del consolidamento fiscale le scelte soprattutto sul versante delle riforme strutturali orientate all'accelerazione del ritmo di crescita, anche usando, sia pure dentro gli spazi limitati di cui ho detto prima, le risorse del bilancio pubblico a fini di sostegno della domanda aggregata, per un verso, e di

I risultati, in particolare nel corso del 2017, sembrano confermare - ripeto - la fecondità di questo approccio. Tutte le scelte compiute nel corso di questi anni e di cui il rendiconto ci fornisce un primo consuntivo sono da considerarsi assolutamente coerenti con questo disegno e quindi da giudicare positivamente? No, non tutte. Quando avremo di fronte

mi auguro che sapremo distinguere tra ciò che ha avuto successo nell'ambito di quelle scelte determinando risultati positivi e ciò che invece si rivela obiettivamente meno efficace e va quindi corretto al fine di un più utile

lo sforzo compiuto per aggredire il problema degli investimenti privati e, con molto meno successo, quello degli investimenti pubblici volti a sostenere il tono competitivo del nostro sistema. Il problema dell'Italia, evidente dai primi anni Novanta, è un andamento insoddisfacente della produttività: sia quella del lavoro sia quella totale dei fattori, cioè lavoro e capitale. A testimonianza che il problema è stato questo, noi durante la grande recessione abbiamo sì avuto una gravissima caduta dei consumi, ma a fronte a fronte della quale nel corso di questi ultimi anni abbiamo realizzato un certo recupero. In termini di dimensioni dei consumi, ormai siamo vicini

il che è un problema enorme perché abbiamo una questione di produttività da risolvere e, se non si fanno investimenti privati e pubblici, la produttività non sale? Nel campo degli investimenti. abbiamo in vigore in questo momento gli incentivi più forti agli investimenti privati, a fini di incremento della produttività, che siano in atto tra tutti i Paesi europei: superammortamento, iperammortamento, credito di imposta automatico per gli investimenti in ricerca, credito d'imposta automatico Sud. Complessivamente, i dati dell'economia reale sembrano testimoniare che questo insieme di risorse funziona. Secondo me sarebbe utile che l'insieme delle forze politiche, al di là della maggioranza e dell'opposizione, volessero constatare la correttezza di questo giudizio, se è corretto; e a me pare che i numeri dimostrino che lo è. Questo al fine di garantire, in un anno preelettorale, gli impegni di tutti a non interrompere questa strada, anche se in un contesto nel quale è evidente che le dimensioni, per esempio, dell'intervento noto come iperammortamento non sono sostenibili nel lungo periodo. È evidente che si tratta di misure straordinarie, volte a recuperare quel gigantesco *gap* che si era aperto nel volume degli investimenti privati nel corso della grande recessione. La caduta è stata superiore al 30 quindi la si recupera solo con misure di carattere straordinario. Le misure di carattere straordinario sono in corso e stanno e stanno funzionando ma dovremo sostituirle con misure di carattere ordinario. Mi fa piacere che prima il senatore Mandelli abbia ricordato il buon funzionamento di una innovazione introdotta quest'anno, cioè i cosiddetti piani di risparmio

allora bisognerà vedere se una quota del risparmio privato saremo stati in grado di orientarla verso l'investimento nel debito delle imprese. Perché questo è un problema strutturale del Paese: il debito delle imprese è troppo concentrato nelle banche e se le banche conoscono una difficoltà, come hanno conosciuto, il finanziamento dell'attività di impresa entra improvvisamente in una situazione vicina al collasso. Sta funzionando la norma sui Piani individuali di risparmio (PIR). Lo spostamento verso gli investimenti in economia reale del risparmio privato italiano è significativo. Quindi, anche a quel proposito dobbiamo cercare norme di consolidamento e impegnarci per un rafforzamento di questa prospettiva ulteriore al di là dell'appuntamento elettorale che ci sarà nella prossima primavera. In questo contesto, naturalmente, hanno fatto bene i relatori a sottolineare questo elemento critico.

Sul versante degli investimenti pubblici, invece, anche negli anni in cui il volume delle risorse stanziate a bilancio è stato superiore a quello dell'anno precedente, in funzione di una accelerazione e di un recupero degli investimenti pubblici, la pubblica amministrazione ha faticato a

Noi possiamo scrivere a bilancio le cifre che vogliamo, ma se non aggrediamo il nodo della concreta realizzazione degli investimenti in termini di procedure, di rapporto tra le amministrazioni, di rapporto tra il sistema della regolazione presidiato dal sistema giudiziario e l'effettiva attività, noi non realizzeremo l'obiettivo di innalzare significativamente, attraverso gli investimenti pubblici, il tono competitivo del Paese. Può darsi che si pensi che questo problema si risolverà da solo mettendo più risorse. Certo, mantenendo lo stesso coefficiente di realizzazione, se le risorse sono di più, vorrà dire che faremo un po' più di investimenti ma resterà il drammatico problema di una pubblica amministrazione italiana che, anche quando sceglie di impegnarsi nella previsione in un volume più significativo di investimenti, non riesce poi a mantenere la promessa implicita in questa scelta. Qui c'è molto lavoro

una volta concluso l'esame degli articoli del rendiconto si passerà direttamente alla discussione degli articoli dell'assestamento. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto congiunte e avranno

l'esigenza di togliere nella parte dispositiva la parola «i», in maniera tale che il testo risulti «per territori interni».